adottata dai colleghi sia di maggioranza sia di minoranza, che tende al ritorno in Commissione dei disegni di legge in titolo, al fine di una trattazione e di un esame approfondito che ne permettano un'analisi e una riflessione tali da evitare scelte affrettate che, evidentemente, nuocerebbero al testo di legge.

vorrei precisare che questi provvedimenti in materia di tortura avevano assunto priorità sia perché il Partito Democratico li ha adottati come propri

a livello internazionale, partendo dalle Organizzazione delle Nazioni Unite fino all'Unione europea. Ricordo che nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva già approvato un provvedimento contro la tortura.

materia fondamentale e importante. Peraltro, va dato atto della necessità di giungere ad un testo unificato, un testo base sul quale lavorare con alcuni emendamenti, in quanto si tratta di individuare la fattispecie giuridica penale più adeguata per combattere il fenomeno della tortura. Vi sono inoltre aspetti che riguardano la giurisdizione, e l'estensione della giurisdizione penale in questa materia. Quindi, siamo d'accordo in merito

Credo però che il percorso che è stato indicato dal senatore Centaro sia quello più corretto. Ci sono diversi disegni di legge che riguardano l'introduzione del reato di tortura, ci sono diverse ipotesi che sono state formulate nei disegni di legge, tuttavia

l'esigenza che il percorso intrapreso non sia lungo. Nel nostro Paese purtroppo si tortura. Nel nostro Paese purtroppo si registrano violenze a più livelli e in più settori. Il nostro Paese rischia di continuare a essere condannato

credo sia interesse di tutti, e del nostro Paese innanzi tutto, non aggiungere troppo tempo alla definizione della materia anche perché, come dicevo poc'anzi, da qui alla prossima primavera il nostro Paese sarà sottoposto ad una verifica relativamente alla qualità dei diritti umani che si garantiscono.

Commissione. **Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano Onorevoli colleghi, con ricorso del 7 aprile 2009 il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali in corso il procedimento penale n. 48698/04 RGNR - n. 20/07 e str. 2345/07 RG GIP, pendente nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 2 novembre 2009, n. 288, depositata in cancelleria il successivo 6 novembre. Nella seduta del 1° dicembre 2009 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituirsi

ha citato varrà, ovviamente, anche per il secondo. Stiamo parlando di conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato. In particolare, il primo che lei ha citato riguarda il caso sollevato dal tribunale di Milano, che ha appunto sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato in relazione alla delibera adottata nella seduta del 19 febbraio 2009 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'ex senatore Raffaele Iannuzzi. Stiamo cioè parlando del fatto se la delibera di insindacabilità adottata dal Senato costituisca o no un'interferenza nelle attribuzioni dell'autonomia giudiziaria, non sussistendo il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare dell'ex senatore Iannuzzi. Siamo cioè oggi chiamati a decidere se il Senato debba costituirsi o no nel giudizio e quindi resistere nel conflitto di attribuzione sollevato. Vorrei ricordare ai colleghi oggi presenti in Aula che sulla questione

alla Camera o al Senato deliberare che i fatti per i quali è in corso un procedimento per diffamazione riguardano o no opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Vorrei solo citare alcune di queste sentenze della Corte costituzionale, che però, come ho detto, costituiscono assolutamente una giurisprudenza

che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti la corte d'appello di Milano un procedimento penale nei confronti di alcuni deputati, per il reato - fra gli altri - anche di diffamazione, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'articolo 68 della Costituzione. sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 4 maggio 2007, in questo caso riguardante un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano in relazione a una delibera del Senato della Repubblica. Anche in questo caso la Corte costituzionale, sempre - lo ripeto - con una decisione conforme, ha ribadito «la piena sindacabilità di dichiarazioni che non costituiscono la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e, quindi, il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (...), ma che rappresentano una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dalla Costituzione E ancora, in questo caso, la Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare per i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del collega senatore. E in ultimo, cito ancora la sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 2007. È evidente quindi, signora Presidente e colleghi, che le pronunce della Corte - per brevità - per brevità ne ho citate soltanto tre, ma posso assicurare, se qualcuno ha la bontà di fare una ricerca, che ve ne sono tantissime altre nella stessa direzione

rispetto all'insindacabilità delle dichiarazioni rese dai parlamentari. Quindi, rimetto all'Aula questa valutazione di carattere più generale sull'opportunità di rivedere la nostra giurisprudenza rispetto a questo tema, anche per non correre il rischio di vederci in continuazione bacchettare dalla Corte costituzionale sul tema.

importante - da parte della Corte costituzionale ad una condanna per lite temeraria. Affido questo ragionamento e questa riflessione all'Aula per il futuro, perché qui ormai una decisione è già stata assunta. Chiedo però all'Assemblea tenuto conto del fatto che verosimilmente anche in questo caso la Corte costituzionale riterrà che il Senato non aveva competenza a pronunciarsi in questa direzione,

Abbiamo deliberato in questa direzione. Ora, sembra che l'Avvocatura dello Stato, nel caso specifico, ritenga non sia il caso di sostenere le ragioni del Senato nel conflitto di attribuzione tra due organismi dello Stato.

del libero Foro che assista e tuteli gli interessi e le ragioni del Senato. Pertanto confermiamo il voto della necessità della costituzione in giudizio. com'è noto, il Gruppo del Partito Democratico non ha ritenuto - né in Giunta delle immunità, nella delibera del 19 febbraio in Aula - che nel merito il caso del senatore Iannuzzi fosse coperto dalla garanzia di insindacabilità delle opinioni dei parlamentari stabilita dall'articolo 68 della Costituzione. Certo, siamo di fronte ad una delibera del Senato che viene portata davanti alla Corte costituzionale per una verifica della sua legittimità costituzionale, cioè del fatto che il Senato, con quella delibera, travalicato i suoi compiti rispetto ai contenuti propri di quella delibera. Riteniamo che il Senato si debba difendere, per un fatto di rappresentazione coerente con quello che a maggioranza esso ha stabilito in quell'occasione. Tuttavia, di fronte alla notizia di una perplessità sulla possibilità di accettare il mandato, per così dire, da parte dell'Avvocatura dello Stato, un pezzo di quella determinazione del Gruppo del Partito Democratico - quello per il quale la causa

Per questo motivo, ci asterremo nella votazione che autorizza il Presidente del Senato alla costituzione davanti alla Corte nel giudizio sul conflitto di attribuzione.

relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Monza - sezione distaccata

si costituisca in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato per resistere nel suddetto conflitto di attribuzione, con l'intesa che se tale proposta non sarà approvata

**Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Monza Sezione distaccata di Desio**

6 novembre. Nella seduta del 1° dicembre 2009 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso all'unanimità nel senso che il Senato debba, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

di spese per il Senato qualora fosse soccombente. In conclusione, confermiamo la stessa indicazione e chiediamo il voto su questa proposizione.

delle immunità parlamentari affinché il Senato si costituisca in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato per resistere nel suddetto conflitto di attribuzione, con l'intesa che se tale proposta non sarà approvata si intenderà accolta la proposta del senatore Izzo di conferire

3 milioni di italiani figurano affetti da questa patologia. Il problema del diabete non è solo la cura

scoprire la malattia prima che essa possa produrre complicanze gravi a carico del nervo ottico, del sistema renale e nervoso. Complicanze assolutamente invalidanti, dalle quali spesso è difficile guarire. Purtroppo, dobbiamo anche dire che, a dispetto del sistema di prevenzione e di cura che il nostro Paese ha istruito, le differenze regionali esistono. Noi, ad esempio, sappiamo che mentre la rete di prevenzione è molto attiva e diffusa nel Nord e nel Centro del Paese, ci sono Regioni del Sud dove la prevenzione avviene solo di nome e non di fatto,

In particolar modo il decreto legislativo n. 124 del 1998 ha riconosciuto il diabete mellito quale patologia invalidante, che dà diritto all'esenzione dal pagamento del *ticket*, tuttavia limitatamente per quelle voci riconosciute nei livelli essenziali di assistenza. Oggi straordinariamente assistiamo al fatto, anche grazie all'evoluzione della tecnica sia diagnostica che terapeutica, molte prestazione connesse alla diagnosi e alla cura del diabete e delle sue complicanze sono escluse dai livelli essenziali di assistenza. Ne consegue che molti pazienti non hanno diritto all'esenzione del *ticket* e devono

addirittura, all'intero delle stesse Regioni, vi si sono differenze nell'ambito delle diverse aziende sanitarie locali. In Lombardia, ad esempio, la fornitura degli *stick* per l'autodiagnosi del diabete

Ma la cosa più grave è che alcune diagnosi e alcuni esami diagnostici per le complicanze non vengono assolutamente esentati. Ad esempio, l'elettromiografia per la diagnosi della neuropatia diabetica periferica - una complicanza estremamente diffusa e grave

invalidante, che ad oggi purtroppo non guarisce nel tempo, ma va trattata dal punto di vista sintomatologico e della prevenzione delle complicanze, molti pazienti si trovano a dover sborsare cifre ingenti - soprattutto per coloro coloro che si trovano in una condizione economica non agiata - per far fronte e curare al meglio la propria patologia. Vi è quindi un problema di prevenzione e di assistenza sul territorio in termini di organizzazione sanitaria, ma anche un problema economico di

dobbiamo muoverci con la coscienza e la responsabilità del legislatore, non fermandoci alla denuncia, ma cercando di intervenire per correggere ciò che non funziona.

presenti in Aula perché dobbiamo condividere insieme la responsabilità per questa patologia importante. Lo faremo sicuramente nella nostra attività politica, nell'impegno che abbiamo nelle associazioni per la prevenzione, ma dobbiamo farlo anche concretamente, garantendo

crisi economica per le famiglie, capite che anche spendere 150-200 euro al mese per una patologia come il diabete è significativo e talvolta crea davvero problemi. Penso che un sistema sanitario solidaristico come il nostro - se la parola «solidarietà» ha un senso e non è

nella Conferenza Stato-Regioni; abbiamo più volte chiesto al Governo di aggiornarci in Commissione sanità sull'andamento di questa discussione, a valle dell'approvazione del nuovo Patto per la salute, che prevede fondi aggiuntivi per il sistema sanitario e le Regioni.

queste prestazioni diagnostiche e questi presidi terapeutici per un'efficace cura e prevenzione del diabete, facendoci carico, vice ministro Fazio - e anche questa è una discussione che abbiamo sempre aperta - di una

Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatori, 3 milioni e mezzo di persone, circa il 6 per cento della popolazione nel nostro Paese, soffrono di diabete.

Mi riferisco alle patologie a carico dell'occhio (quali la retinopatia) o del rene, a forme di patologia a carico dell'emuntorio renale che determinano anche il ricorso alla dialisi e al trapianto. dimentichiamo i problemi relativi al piede diabetico, che determinano, in una percentuale elevatissima di casi, anche amputazioni. Ancora, solo il 15 per cento della popolazione diabetica - secondo dati provenienti da fonti assolutamente accreditate

Ogni anno la popolazione diabetica aumenta di circa 150.000 unità. Il diabete è la quarta causa di morte del nostro Paese: 18.000 persone - secondo dati ISTAT - ogni anno muoiono per la patologia diabetica. Queste sono le motivazioni per le quali il diabete è una patologia sociale. È una patologia sociale che trova attento il Governo, che trova attente la comunità scientifica, le società rappresentative dei pazienti diabetici. Questo è il motivo per il quale nel nostro Paese, ormai dal 2001, si celebra la Giornata del diabete, che trova uno straordinario momento di testimonianza solidale e civile

termini complessivi le sinergie di tutto un mondo che guarda con attenzione ed apprensione a questo problema. Le iniziative si si celebrano ogni anno e sono finalizzate a far crescere l'attenzione nella nostra comunità e a sensibilizzare anche la parte politica a livello sia nazionale che regionale. Che il problema sia allarmante lo dimostra anche il fatto che nel 2006, con la risoluzione 61/225, l'Assemblea generale dell'ONU ha stabilito che

e per il mondo intero. Si consideri che in Italia il 7 per cento della spesa sanitaria generale viene destinato alla terapia e alle cure per il diabete, e parliamo di circa 6 miliardi di euro. quindi, che l'iniziativa di condividere la mozione presentata dalla collega Baio e da altri colleghi, sottoscritta in modo condiviso da maggioranza e opposizione, sia il gesto più maturo e responsabile di un impegno che ci vede congiuntamente protesi protesi verso l'individuazione dei punti di criticità che devono formare l'oggetto della nostra richiesta al Governo di proseguire nella direzione che già con particolare concretezza viene realizzata, lasciando lasciando impregiudicati anche su questo versante quei princìpi che fanno forte il nostro Sistema sanitario nazionale e che sono ispirati alla solidarietà, alla omogeneità

fondamentale principio del solidarismo e della omogeneità dei trattamenti, indipendentemente dalle condizioni

devono introdurre in sede di rielaborazione dei livelli essenziali di assistenza tutte quelle prestazioni che afferiscono alla patologia diabetica in modo diretto,

creare le condizioni affinché il paziente diabetico possa svolgere una buona attività di monitoraggio attraverso una costante e periodica misurazione misurazione della glicemia, cosa che poi determina una corretta posologia nella somministrazione dei farmaci.

complicanze determinate dal cosiddetto piede diabetico: in Italia vi sono circa 6.850 amputazioni derivanti dal piede diabetico, che generano circa 150.000 giornate di degenza; solo per il piede diabetico si spendono 81 milioni di euro. Pertanto, intervenendo in questa direzione, non soltanto creiamo una condizione di omogeneità,

corretto accesso in termini di gratuità alle prestazioni del servizio sanitario nazionale: ciò rappresenta un atto di civiltà e di attenzione verso una patologia

costi sociali indotti. Al riguardo ho molto apprezzato l'impegno del Governo ed, in particolare, del vice ministro Fazio quando in più occasioni, da ultimo a Ferrara nello scorso mese di novembre, evidenziato come nell'ambito delle attività di prevenzione debba essere inserita anche quella fisica come farmaco. Questo è un passaggio straordinariamente importante

delle condivise indicazioni di impegno che rivolgiamo al Governo possa trovare riscontro positivo anche in una sanità equa, solidale e orientata ai principi dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza.

È la sfida del nostro Paese, di noi politici. So che spesso si preferisce la cura diretta alla spesa in farmacia o altro, ma questa rivoluzione culturale (che comporta una educazione continua) parte dalla scuola,

Caro Vice Ministro, questo è uno dei temi classici nei quali si riscontra che il sistema sanitario è un crocevia tra sviluppo del Paese, e quindi investimenti,

a questo nostro Parlamento che rappresenta gli interessi di tutti gli italiani e al nostro Governo dobbiamo ricordare strumenti che aiutino a interagire con le Regioni, senza consentire però a queste ultime di tirarsi da parte per motivi organizzativi e finanziari. La situazione attuale del sistema sanitario dal punto di vista finanziario ci è nota; ci addolora che ci siano Regioni commissariate. È curioso d'altra parte che vengano commissariate con i Presidenti a testimonianza che c'è qualcosa che non torna perché le responsabilità devono essere diversificate: il Presidente di una Regione deve essere votato, il commissario deve rappresentare gli interessi generali del Paese e del Governo. Il diabete è tutto ciò che è stato detto poco fa, ma la prevenzione, e quindi la conoscenza anticipata del rischio di malattia, è il problema. problema. Abbiamo bisogno di un'attenzione da parte di tutti i professionisti, perché il diabetico oltre ad avere il suo medico di famiglia, qualche volta deve rivolgersi ad un oculista,

LEA. Il progetto obiettivo supera quella ristrettezza di dibattito che rimane chiusa nella Conferenza Stato‑Regioni. Questo è un argomento che forse ieri, durante la discussione delle mozioni sulle riforme, avremmo potuto citare perché se quest'Assemblea diventasse il Parlamento delle Regioni forse di questo parleremmo. Se se ne parla solo nella Conferenza Stato‑ Regioni nel momento in cui dibatte contrattare la divisione del fondo sanitario regionale, questi temi non diventano di dominio comune e non ci si accorge che questo Parlamento si sta interessando ai bisogni veri

pensioni di invalidità avremmo, cittadini che continuano a lavorare che non sarebbero invalidi, che non subirebbero alcuna amputazione: la dignità e l'integrità della persona a fronte di operatori che sappiano fare il loro lavoro e che riconoscono prima prima il rischio e poi l'evidenza di questa malattia. Mi sono permessa di presentare un disegno di legge che credo i colleghi potranno esaminare con una certa attenzione, perché uno dei problemi grossi è il piede diabetico. Allora, invece che affidarsi ai pedicuristi o ad altri che fanno un lavoro magnifico dal punto di vista estetico, bisognerà magari dedicarsi, come nel resto d'Europa, in Spagna per esempio, o come negli Stati Uniti da molto tempo o in Australia, al podologo, professione sanitaria e non medica, che non medicalizza - quindi costa di meno ma fa un lavoro particolarmente adatto alla cura del piede diabetico e impedisce quindi un'eventuale amputazione. Abbiamo a che fare con questo crocevia di organizzazione sanitaria,

una nuova tappa importante. Incominciammo con i centri di riferimento regionali e arriveremo forse ad una programmazione nazionale che valorizza anche il ruolo delle Regioni ma che dà giustamente al Parlamento e al Governo l'opportunità di pensare all'intero Paese.

Siamo stati mossi particolarmente da una preoccupazione, cioè la forte diffusione che ormai ha questa malattia. Tra l'altro, leggendo il rapporto annuale, che ormai viene pubblicato regolarmente a livello mondiale dal 2007 e raccoglie tutte le informazioni sull'andamento della lotta contro il diabete, i dati sono veramente allarmanti. Prima di tutto si registra l'aumento di questa malattia sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, e questa dei Paesi in via di sviluppo, ad esempio, è una novità; ma il peggio, anche secondo i dati della Federazione internazionale del diabete, deve ancora venire. Si prevede infatti che nel 2025 saranno 380 milioni le persone malate di diabete nel mondo. Le ragioni di questo *trend* sono legate principalmente all'invecchiamento della popolazione, però anche all'aumento dell'obesità, forse questa sarebbe una delle preoccupazioni che dovremmo avere riguardo alla definizione di un piano di prevenzione più generale,

e, secondo alcuni dati, questa spesa dovrebbe passare da 132 miliardi di euro del 2002 ai 192 miliardi nel 2020. In Italia, nel 2006, si calcola che il 4,5 per cento della popolazione abbia avuto un trattamento per il diabete, con un aumento di quasi dieci punti rispetto a dieci anni fa, quando eravamo al 3,1 per cento. Di fronte a questi dati è chiaro che tagliare i costi del trattamento non è assolutamente la soluzione, perché questo poi vuol dire che saranno di gran lunga maggiori i costi del trattamento delle complicanze e delle conseguenze che questa malattia porta con sé. Quindi, è solo grazie ad una buona prevenzione, alla diagnosi fatta il più tempestivamente possibile, ad un'efficace gestione e cura della malattia che si possono evitare tali complicanze e quindi la la possibilità di mantenere a chi è malato una certa qualità della vita. Occorrono quindi degli interventi educativi, che oggi mancano, occorre una vera e propria alleanza tra gli operatori sanitari e i pazienti per poter gestire nel tempo una malattia che è cronica e quindi si protrae per molti anni lungo l'arco della vita delle persone che si ammalano. Vorrei anche ricordare che in Italia, dal punto di vista legislativo, siamo stati all'avanguardia rispetto alle necessità di cura di questa malattia. La legge n. 115 del 1987, infatti, istituiva già allora

dagli specialisti che operano in questi centri; l'altro 40 per cento però è seguito dai medici di medicina generale o non si cura. anche sulla base dell'esperienza realizzata in questi anni, molti medici di medicina generale denunciano la difficoltà con questi centri rispetto alle esigenze dei propri pazienti e anche la difficoltà di avere un ritorno rispetto a come questi pazienti vengono curati nei centri. Quindi, vi è l'esigenza di creare una rete sul territorio che consenta ai medici di medicina generale ed a tutti gli operatori dei servizi che riguardano malattie di tipo cronico come questa, una reale possibilità di comunicazione, che sarebbe produttiva per tutti, ma in particolare per i pazienti. Non possiamo non riconoscere che in questi anni gli operatori sanitari, il volontariato, l'associazionismo professionale sono stati veramente preziosi e dobbiamo anche dire che molte Regioni si sono mosse in maniera estremamente utile e positiva per far fronte a questa malattia e alla sua diffusione. Non possiamo però neanche nasconderci che l'esistenza di grosse differenze di grosse differenze tra Regioni comporta il fatto che nel nostro Paese la prevenzione e la cura del diabete si svolgano in modo diverso e quindi determinino in maniera concreta una diversa accessibilità al diritto alla salute da parte dei nostri cittadini. È quindi necessario intensificare l'iniziativa, anche in rapporto all'appello dell'ONU che, nel dicembre 2006, dall'Assemblea generale ha lanciato un richiamo a tutti gli Stati membri perché in tempi rapidi vengano presi provvedimenti che vadano nella direzione dello sviluppo di politiche nazionali di prevenzione e trattamento della cura del diabete. La risoluzione dell'ONU prende proprio le mosse dal riconoscimento del diabete come malattia cronica che ha delle complicanze molto gravose e che incide pesantemente, non solo dal punto di vista umano, ma anche sul piano economico. Cruciale per questo diventa la difesa e l'implementazione della salute pubblica attraverso adeguati interventi di assistenza sanitaria. Gli studi condotti in questi anni hanno dimostrato che investire in prevenzione e in cure efficaci comporta un notevole risparmio in termini di disabilità e di sofferenze, nonché di costi diretti e indiretti per la cura delle complicanze. origine il senso che viene dato alla nostra mozione; chiediamo appunto al Governo un impegno particolare perché oggi diverse prestazioni, sia per la prevenzione che per la cura, non sono incluse nei livelli essenziali di assistenza. Ad esempio, veniva riportato che i presìdi per l'autocontrollo della glicemia vengono concessi in modo differenziato e carente dal Servizio sanitario nazionale;

Conosciamo tutti le problematiche legate al rinnovo dei livelli essenziali di assistenza, che sono stati bloccati nel 2008 perché si è detto che non vi erano risorse sufficienti;

quello che chiediamo tutti, anche in modo *bipartisan*, è l'accesso alle cure e alle prestazioni per i pazienti diabetici su tutto il territorio nazionale (eliminando quindi le differenze che oggi ci sono) e la gratuità delle prestazioni connesse alla cura del diabete. Ci auguriamo quindi che la discussione che oggi si svolge in quest'Aula, autorevole ancorché purtroppo poco frequentata, non sia solo un atto di attenzione a questa grave malattia che interessa circa 45 persone ogni mille abitanti, ma sia anche l'occasione per dare una risposta concreta a questi malati, al loro bisogno di cura, alle loro famiglie e sia anche l'occasione per dare il via a un vero e proprio piano di prevenzione generale per il nostro Paese. *(Applausi finestra"). Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del liceo classico "Gorgia" di Lentini, Siracusa, ai quali diamo il benvenuto. Signora Presidente, visti i pochi minuti a disposizione chiedo sinteticamente di poter aggiungere la mia firma a questa mozione e di poterla arricchire con un impegno nei confronti del Governo a potenziare l'educazione sanitaria nelle scuole per prevenire tutti i fattori di rischio che stanno portando i nostri giovani precocemente incontro al diabete. Chiedo, in secondo luogo, di inserire nella mozione un appoggio all'iniziativa del vice ministro di promuovere una vera attività fisica, non solo nelle scuole ma anche successivamente, per favorire la prevenzione nei confronti di tante malattie e in particolar modo del diabete. Invece di ripetere quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto e che condivido, vi racconto un aneddoto. Nei giorni scorsi,

per la vendita di merendine e soda, bevande altamente glicemiche che danno tanto zucchero ai nostri giovani. La signora, madre di tale Roberto, dopo poche ore scopre che il figlio obeso ha il diabete, a otto anni e, guarda caso, avrebbe dovuto sapere che le merendine che verranno vietate in California sono una delle maggiori cause di diabete per i nostri giovani, insieme alla scarsa attività. Inoltre, avrebbe già obeso a otto anni, senza praticare la ginnastica, è andato incontro più facilmente dei suoi coetanei al diabete e probabilmente a 40 anni avrà già

questa affermazione. Se non avremo il coraggio di intervenire come Parlamento, come Governo, indipendentemente da maggioranza e opposizione, senza giocare sulle parole, probabilmente non verremo rispettati dai nostri cittadini.

osservo quanto segue. Nel merito del primo impegno posto, il diritto alle cure viene garantito ai malati con diabete, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza così come avviene per altri pazienti con altre patologie. In particolare, per quanto riguarda l'accesso omogeneo alle cure per i pazienti diabetici su tutto il territorio nazionale, posso confermare che tutte le Regioni sono attualmente coinvolte nello sforzo di riorganizzazione e razionalizzazione dell'assistenza diabetologica in Italia e il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2010-2012, in via di perfezionamento, dovrà rinnovare gli obiettivi proposti dal precedente piano in modo da consentirne il raggiungimento. Com'è noto, il piano prevede un livello di prevenzione primaria degli stili di vita, in cui si include anche l'attività fisica e il controllo dell'alimentazione; un livello di prevenzione secondaria della popolazione a rischio, cioè di chi ha già sviluppato dei fattori di rischio; un livello di prevenzione terziaria, che è la prevenzione delle recidive nella popolazione che ha già sviluppato la malattia. Ricordo che, al fine di sostenere e coordinare i progetti regionali afferenti al Piano nazionale della prevenzione (PNP), già dal 2006 (ma è tuttora operativo) il progetto IGEA del Centro di controllo delle malattie (CCM), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, ha avuto il compito di

le aziende unità sanitarie locali, provvedano a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura, i presìdi diagnostici e terapeutici di cui al decreto del Ministro della sanità

reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glucosemia - test rapido con una goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso), anche i riflettometri per la lettura rapida della glicemia, i microinfusori per l'infusione programmata dell'insulina, nonché gli altri mezzi meccanici per l'erogazione dell'insulina e tutti gli strumenti utili per il trattamento del diabete. L'individuazione della malattia diabetica fra le condizioni di malattia croniche e invalidanti garantisce a questi pazienti, in esenzione dalla quota di partecipazione, l'utilizzo di prestazioni specialistiche ambulatoriali appropriate, come da decreto legislativo n. 124 del 1998. Inoltre il Ministero, nell'ambito dei nuovi LEA, ha provveduto ad aggiornare il «pacchetto prestazionale» garantito ai diabetici, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale per la malattia diabetica, la scelta degli accertamenti erogabili in esenzione è stata condivisa con le società scientifiche e le associazioni dei pazienti, nel rispetto dell'appropriatezza assistenziale e ai fini del monitoraggio della patologia, della prevenzione delle complicanze, del monitoraggio degli effetti collaterali della terapia farmacologia e del *follow up* delle eventuali patologie associate, nell'ambito appunto del progetto di prevenzione terziaria. Tra le prestazioni inserite, confermo che sono presenti quelle utili per la gestione della neuropatia diabetica e del piede diabetico, quelle finalizzate all'autocontrollo (educazione terapeutica) ed altre mirate a tutelare più efficacemente il soggetto con diabete (per esempio, monitoraggio dinamico

ringrazio il Vice Ministro, che ha accolto questa mozione, ma vorrei *in primis* ringraziare la senatrice Baio, che con grande sensibilità ha posto all'attenzione della nostra Aula questa problematica.

ma ha bisogno di essere curato con attenzione e anche con molto rispetto; un rispetto che normalmente ci facciamo mancare, proprio perché non ci vogliamo bene e quindi mettiamo in campo noi stessi delle controazioni che poi

stratosferici, enormi, e quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di controllare, di verificare, di attuare una particolare forma di monitoraggio, perché

dopo queste grandi discussioni, ha deciso e ha vinto la sua battaglia, tant'è che non fuma più, e di questo siamo tutti contenti.

Visto che l'uomo è fatto per vivere e ognuno di noi vorrebbe che la propria morte fosse il più lontano possibile, riflettiamo su questo e diciamo ai nostri concittadini che il diabete è una fonte di diminuzione della vita personale. Per questo abbiamo assolutamente bisogno - ritorno qui alla prima parte del mio intervento - di volerci più bene, di controllarci maggiormente e di avere stili di vita più corretti.

Sicuramente in questa battaglia contro questa epidemia un grande spazio va dato all'informazione. Un'informazione che deve rivolgersi anche all'obesità e ai disturbi alimentari, soprattutto alla cattiva alimentazione.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, il Gruppo dell'Italia dei Valori vuole confermare e rafforzare con piena convinzione

in modo particolare all'autorevolezza del Vice Ministro - senza polemica, perché questa mattina in Aula si è trovato un momento di ampia e forte condivisione su un tema, affrontato da autorevoli relatori che mi hanno preceduto, di grande importanza sociale.

approfittando forse di uno spazio di riserva, di un'area di risulta dell'attività parlamentare, in quanto siamo in attesa del ritorno della finanziaria dalla Camera dei deputati. Diciamoci le cose senza siamo in attesa della finanziaria di ritorno dalla Camera dei deputati e che decolli il processo breve e, quindi, in questo spazio morto dell'attività parlamentare, parliamo di un problema straordinario che interessa 3 milioni di italiani. Vorrei che questo dato cronologico fosse solo una coincidenza; come medico e come italiano, voglio illudermi che sia soltanto questione di coincidenza. Vengo alla seconda considerazione, signora Presidente. sembra assurdo considerando gli effetti importanti che questa mozione ha saputo ripresentare all'attività dell'Aula,

temi semplici: la mozione chiede la gratuità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche su una malattia sociale di grande rilevanza e l'uniformità in tutte le Regioni d'Italia. Allora, su questi due punti, l'altra considerazione

vi era anche la necessità di una distribuzione gratuita dei fondamentali presidi diagnostici e terapeutici. È evidente che dal 1987 le conoscenze scientifico-mediche sono notevolmente mutate. Era altrettanto evidente che l'adeguamento da parte di un Servizio sanitario nazionale pubblico a questi miglioramenti delle conoscenze tecnico-scientifiche dovesse essere necessariamente un atto dovuto,

distinguendoli tra permessi brevi e permessi per malattia; chi matura un certo numero di giorni per malattia non ha più diritto a premi di produzione e a quant'altro. Il malato diabetico mi ha

buone intenzioni di una adeguata prevenzione e terapia del diabete, si deve sottoporre a trattamenti presentandoli come malattia e quindi, come tale, è discriminato sul posto di lavoro.

di cultura, di come noi affrontiamo patologie del genere che sono di grande rilevanza sociale. Non dobbiamo scimmiottare i Paesi anglosassoni o i Paesi esteri.

individua alcuni metodi di approccio del cittadino diabetico nei confronti di questa patologia invalidante.

Sarà per nostra deformazione professionale di Gruppo senatoriale, ma l'aspetto che più ci piace è il bellissimo richiamo fatto nella mozione

vengano garantiti tutti i presidi diagnostici, anche alla luce delle moderne acquisizioni e conoscenze scientifiche.

riferimento come punto importante. Da tale studio risulta che dalla Basilicata all'Umbria fino alla Lombardia vi sono comportamenti, trattamenti, assistenze, servizi e strutture completamente diversi.

un livello minimo ed essenziale per i cittadini affetti da tale patologia.

che ha voluto sottolineare un principio fondamentale di educazione sanitaria, partendo dalle scuole e dai ragazzi. La vera sfida

interventi. Concludo rafforzando un concetto che non è emerso, se non in maniera molto velata, nel dibattito di questa mattina. I centri di diabetologia sono sicuramente importanti: rappresentano punti di riferimento sul territorio, sono fortunatamente tanti e distribuiti su tutto il territorio nazionale e svolgono un ottimo lavoro.

che tanti arti salvano e che tanta prevenzione possono favorire nel caso di piede diabetico. Le camere iperbariche, molto spesso demonizzate, ma sicuramente troppo poco presenti sul nostro territorio, rappresentano un'ulteriore possibilità di migliorare in maniera decisiva la vascolarizzazione degli arti dei diabetici, ma non vi si fa quasi mai ricorso perché ce ne sono poche, sono scomode, costano e non vengono convenzionate con i centri. Per questo mi sento di stimolare il

ma l'influenza non determina le invalidità che può determinare il diabete, e 250 milioni di individui affetti in un anno costituiscono una vera e propria pandemia. Credo che l'allarme sanitario debba suonare, gli scudi debbano alzarsi, ma soprattutto tutte le armi a disposizione debbano essere messe in campo.

La mozione che stiamo per votare è una scelta importante per i pazienti diabetici, per le loro famiglie, per le associazioni che si occupano di queste persone e per l'intera società.

che un paziente diabetico ha, soprattutto quando vede negati alcuni dei suoi diritti. La scelta che stiamo facendo oggi è quindi un atto di civiltà,

Come è stato ricordato, i diabetici rappresentano oggi circa il 4,5 per cento della popolazione, pari a circa 2,6 milioni di persone, ma si stima che in Italia i malati siano 3,5 milioni, pari al 6 per cento della popolazione. significa che quasi un milione di persone è affetto da questa malattia, ma non sa di essere malato; sta male, ma non sa di cosa, anche perché alcune volte si fatica a fare la diagnosi; non è quindi sottoposto ad alcun trattamento. Si stima che entro il 2010 in Italia si arriverà a 4,5 milioni di persone

affinché possa curarsi adeguatamente attraverso un autocontrollo, che è l'elemento essenziale per i pazienti diabetici. Serve un sistema sanitario che sappia andare incontro al malato, serve l'aspetto diagnostico, così come l'aspetto terapeutico, ma l'autocontrollo, per un malato cronico,

D'altro canto, il diabete è una pandemia sociale maledettamente silente; se si manifestasse in modo più evidente, sarebbe più semplice da diagnosticare e da curare. Invece - uso questo termine volutamente - è maledettamente silente.

purtroppo - non vorremmo dirlo, ma è così - esiste una discrepanza nell'applicazione della legge sia tra le diverse Regioni sia all'interno delle stesse Regioni. Occorre quindi un controllo maggiore da

non si manifestano in modo evidente. Certo, un professionista esperto, un medico, le sa diagnosticare bene: lei lo sa, professor Fazio, perché viene da una delle maggiori cliniche diabetologiche presenti sul territorio nazionale. Purtroppo, però, non sempre il paziente diabetico incrocia il il professionista serio, come diceva prima anche il collega Mascitelli. Voglio portare un esempio - che è già stato citato - per far capire di cosa stiamo parlando e perché abbiamo scritto e condiviso questa mozione.

La logica del reale bisogno del paziente, però, non è presente su tutto il territorio nazionale, perché purtroppo prevale la logica dell'economia della Regione di riferimento. Lo dico abbassando il tono di voce: non ce l'ho con nessuno, però non si può negare ad un paziente diabetico la striscia per la rilevazione della glicemia: sembra che ogni volta debba dimostrare di essere diabetico e debba farlo chiedendo la carità.

tutte le leggi e tutte le dinamiche organizzative del sistema sanitario nazionale, si vede negato il suo diritto. Tra le tante persone che mi hanno scritto,

dei pazienti che prendono gli ipoglicemizzanti. Questo signore, come tanti altri, si sente incompreso nella gestione della sua malattia, e di conseguenza abbandonato. Come dargli torto? Il paziente diabetico, affetto da una cronicità che in alcuni casi dura un'intera vita, si trova spesso a dover giustificare la sua malattia; deve spesso dimostrare di esserne affetto per vedersi riconoscere almeno una parte dei suoi diritti.

alcune prestazioni relative a complicanze connesse al diabete sono addirittura escluse dai LEA. In particolar modo vorrei soffermarmi sul cosiddetto piede diabetico, che incide sul 4-5 per

i dati ci fotografano una realtà agghiacciante: la prevalenza di amputazioni totali equivale al 3,6 per cento su 100.000 casi, ovvero in Italia il numero di amputazioni è pari a 6.197, di cui 2.067 sono amputazioni maggiori: riguardano la gamba, cento dei diabetici che ha un'ulcera ad un piede andrà incontro ad un'amputazione; il 50 per cento degli amputati subirà entro cinque anni una seconda amputazione; cento degli amputati ha un elevato rischio di morte entro cinque anni. I danni psicologici, oltre che fisici, sono inestimabili. Il nomenclatore tariffario nazionale, non aggiornato da un decennio, ad oggi prevede che i pazienti con piede a rischio per

che vengono cambiate soltanto qualora usurate. Inoltre, non essendo aggiornato, non permette una corretta valorizzazione economica dei presidi oggi disponibili sul mercato. La maggior parte della persone affette da piede diabetico è anziana, di conseguenza passa la maggior parte del tempo in casa: ha pertanto necessità di disporre di una ciabatta o di un sandalo. Mi spiace dire queste cose, ma lo faccio per far capire la banalità la banalità di quello che manca in Italia. Abbiamo una buona legge, che prevede dei benefici, eppure, maledettamente, queste persone sapete a cosa sono sottoposte? A dover chiedere l'invalidità, perché altrimenti questi non vengono loro riconosciuti. Ma perché mai una persona deve dire di essere invalida, quando non lo è?

decisamente riprendere in mano il problema e affrontarlo nella sua interezza. Vogliamo correggere queste storture applicative perché sono un nonsenso, e nessuno di noi pensa di voler realizzare un nonsenso, almeno, sicuramente, noi che siamo qui. Approvando questa mozione, e con la volontà del Governo, possiamo davvero dare una risposta concreta al diabetico e cerchiamo di farlo mutuando le esperienze delle Regioni che oggi fanno di più e meglio rispetto ad altre.

Accanto a questo, oggi permettiamo anche l'applicazione di una dichiarazione scritta presentata e approvata dal Parlamento europeo

potranno, speriamo, vivere meglio. Noi come Parlamento ci impegniamo a essere vigili, e lo faremo trasversalmente. Saremo vigili affinché quanto è stato detto oggi in questa sede diventi vita vissuta per tutti i pazienti diabetici. Sono certa che che già questo pomeriggio queste persone ringrazieranno il Governo e tutti noi.

Non vorrei infatti che qualcuno si facesse bello in televisione dicendo che tutto va bene, quando questo servizio non viene assicurato nei giorni di festa. Capisco che questo problema apparire minore, ma non tanto, perché chiunque, che sia temporaneamente senatore o parlamentare o semplice cittadino per tutta la vita, può constatare che sulle autostrade italiane quel servizio non funziona,

Signor Presidente, nel dicembre 2008 il Ministro dell'interno, in attuazione della legge sulla contabilità pubblica degli enti locali, ha sciolto il Consiglio comunale del Comune di Capistrello, in provincia dell'Aquila, e ha correttamente nominato un commissario straordinario pochi mesi dopo (due o tre), attraverso un compendio molto elaborato di numerose decine di pagine, ha dichiarato con un proprio provvedimento il dissesto finanziario di quel Comune. Lei mi insegna quali sono le procedure derivanti dal dissesto finanziario, cosa comporta sugli organi che successivamente verranno eletti e quali sono i riflessi sulle popolazioni dei Comuni nei quali è stata dichiarata tale procedura. Risulta agli atti del Senato che nel corso dell'anno 2007, con provvedimenti amministrativi di questa Camera, il suddetto Comune ha beneficiato di numerose centinaia di migliaia di euro per la realizzazione di opere in conto capitale. Di questi denari, con atti amministrativi correttamente formulati e comunicati con decreto del Ministro dell'economia, non vi è traccia all'interno dei provvedimenti sul dissesto finanziario. Con lettera dello scrivente, signor Presidente, allegando tutti gli atti legislativi, normativi e amministrativi, è stata chiesto al commissario straordinario di riferire che fine avessero fatto questi soldi.

non ha mai risposto, salvo inviare allo scrivente una lettera, verso la metà di ottobre, in cui si diceva che gli uffici stavano predisponendo la risposta.

presso il Ministro dell'interno affinché solleciti, nelle forme e nei modi consentiti dall'ordinamento vigente, il commissario straordinario del Comune di Capistrello a rispondere

Senatore Lusi, la risposta è quasi impossibile, perché non esiste una modalità di intervento informale.

è proprio a tutela del parlamentare; diversamente ci si affiderebbe al buon cuore del Presidente di turno. In una democrazia, però, non ha senso affidarsi al buon cuore: affidiamoci alle regole.